Signor Presidente, è morto qualche giorno addietro Francesco Forte. Se n'è andato in punta di piedi, nei giorni peggiori, quelli delle feste, ammesso che ce ne siano di migliori. Francesco Forte è stato parlamentare, nostro collega dal 1987 al 1994, eletto nelle file del Partito Socialista, fino alla sua distruzione per mano giudiziaria. Un'intelligenza lucida fino agli ultimi giorni della sua vita, cui spesso in questi anni molti appartenenti alla mia area politica hanno attinto. Un instancabile pedagogo. Ricordo certe notti, quando lui, già in età avanzata, a me esausta continuava a dispensare perle di saggezza, lucide analisi, consigli preziosi, ma soprattutto umanità. Economista di vaglia, più volte ministro e sottosegretario per il Partito Socialista; era un intellettuale a tutto tondo e un vero socialista liberale. Per lui la libertà era un valore non negoziabile era un gran sostegno sia verso chi esprimeva un talento, sia verso chi mostrava un bisogno. Detestava chi pensava di avere la verità in tasca ed era lui stesso un uomo libero e un *hombre vertical*, come si direbbe in Spagna. È stata una figura largamente sottovalutata. Se non fosse stato un socialista craxiano, un compagno leale, nella buona e nella cattiva sorte, anche nella "seconda Repubblica" avrebbe avuto altri incarichi e alla sua morte gli sarebbero stati tributati ben altri onori.

Infatti, ricordo che proprio Bettino, dopo l'esperienza di Governo alla guida dei dicasteri dell'economia, prima, e delle politiche comunitarie, dopo, lo volle Sottosegretario delegato per gli interventi straordinari del Terzo mondo nel suo secondo Governo, rafforzando ancora di più un sodalizio che, prima ancora che politico, era umano. Tale comunanza di visioni continuò negli anni in cui Craxi svolse l'incarico di rappresentante personale per il Segretario generale dell'ONU, Javier Pérez de Cuéllar, per l'abbattimento dei debiti del Terzo mondo. Francesco, con i suoi studi, fu un valido collaboratore per mettere a punto quel piano di riscatto e di dignità ancora oggi di straordinaria attualità. Lo voglio salutare qui, chiedendo all'Assemblea di ricordarlo con un minuto di silenzio. Lo voglio salutare come si fa tra compagni socialisti: ciao, Francesco.

Gli emendamenti sono stati presentati col termine, non prorogato, del 14 dicembre. Da allora sono passati giorni e ancora non si è potuto iniziare l'esame degli emendamenti, perché nell'ambito della maggioranza ci si deve mettere d'accordo. Dovevamo iniziare i lavori alle ore

si trovava nel corridoio, fuori dall'aula della Commissione. La Costituzione e la decenza dicono che le leggi si discutono in Aula o in Commissione, davanti ai cittadini, con un verbale e non in interminabili negoziati nell'ambito della maggioranza o nell'ambito di chi chi volete voi. Questo va benissimo, è normale che succeda, ma bisognerebbe rispettare un minimo di decenza nei tempi, perché questi provvedimenti incidono pesantissimamente sulla vita degli italiani e non possono essere discussi nei corridoi, italiani e non possono essere discussi nei corridoi, a scapito totale della possibilità di esaminarli dove si può votare, dove la Costituzione stabilisce che si debba votare e cioè in Commissione e in Aula. Non sfugge

arriva nelle sedi proprie, istituzionali, in una situazione nella quale per di più esaminiamo un decreto-legge che è stato ampiamente superato da tutti gli altri, se non per alcuni dettagli, sui quali comunque riescono a

una nuova finestra"). In base alla deliberazione adottata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 16 dicembre 2021, comunicata dal Presidente della Giunta medesima in data 20 dicembre 2021, occorrendo provvedere all'attribuzione del seggio resosi vacante nella circoscrizione estero, ripartizione America meridionale, il senatore subentrante è il dottor Fabio Porta. Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari della comunicazione e proclamo senatore Fabio Porta. Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Presidente, in queste ultime tre ore abbiamo fatto più di 100 votazioni degli emendamenti al decreto-legge, però non siamo stati in grado di terminare l'esame del provvedimento. Ci manca ancora qualche voto, per il quale avremmo bisogno di altre due ore di tempo.

scusate per questa immissione fuori campo, ma abbiamo appena saputo che la Commissione bilancio ha bisogno di un'altra mezz'ora

lo scioglimento della riserva da parte della Commissione bilancio sugli ultimi nove emendamenti, sono costretto a chiederle un ulteriore rinvio. Dopo aver sentito il presidente Pesco,

preventivamente restringere i tempi di discussione dei singoli senatori (naturalmente l'Assemblea è sovrana),

Signor Presidente, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, reca misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il provvedimento si compone di 10 articoli, suddivisi in tre capi. Nell'ambito del capo I, l'articolo 1 novella il decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di modificare la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgano la loro attività nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie o parafarmacie e negli studi professionali e per i lavoratori anche esterni, operanti a qualsiasi titolo in strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, *hospice*, strutture riabilitative, strutture residenziali per anziani, strutture socio-assistenziali, semiresidenziali e strutture che a qualsiasi titolo ospitino persone in situazioni di fragilità. In primo luogo si specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame. Si sopprime il termine del 31 dicembre 2021, finora vigente per gli obblighi in esame. *(Brusìo. Richiami del Presidente).* Resta ferma l'esenzione, permanente o temporanea, per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione in oggetto. Per gli esercenti una professione sanitaria, il controllo dell'adempimento dell'obbligo vaccinale è demandato agli ordini professionali, mediante verifica dei certificati verdi Covid-19 ed è confermato il principio della sospensione da ogni attività lavorativa per il caso di inadempimento. Per gli altri lavoratori in ambito sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto-legge. L'articolo 2 reca anch'esso modifiche al decreto-legge n. 44 del 2021. In particolare, prevede che l'obbligo vaccinale sia esteso a decorrere dal 15 dicembre 2021 alle seguenti categorie: personale scolastico del sistema nazionale d'istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che organizzano percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore; personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale nonché personale del Dipartimento delle e sicurezza interna. Si dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa e che i dirigenti scolastici e gli altri responsabili delle istituzioni in cui presta servizio il suddetto personale assicurino il rispetto e l'obbligo vaccinale. Si rendono altresì applicabili disposizioni di cui all'articolo 1 del presente decreto concernente i soggetti esenti dall'obbligo vaccinale. Si definisce la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa senza retribuzione per non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Per la sostituzione del personale scolastico che non ha adempiuto all'obbligo vaccinale sono attribuiti contratti a tempo determinato, che si risolvono di diritto nel momento nel quale i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa. Infine, sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento di attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali anche per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti. Il capo II riguarda, invece, l'impiego delle certificazioni verdi Covid-19. In particolare, l'articolo 3 novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 integrando integrando a decorrere dal 15 dicembre dello scorso anno la disciplina delle certificazioni verdi Covid-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successivo al completamento del ciclo vaccinale primario. Inoltre, riduce, sempre con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione o dall'eventuale dose unica prevista e specifica per il medesimo periodo di validità, che decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo. Anche l'articolo 4 introduce modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021 con decorrenza dal 6 dicembre 2021. Nello specifico, modifica l'articolo 9-*bis* relativo all'impiego di certificazioni verdi Covid-19 inserendo gli alberghi e le altre strutture ricettive tra le attività per usufruire delle quali è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi. Conseguentemente non fanno più eccezioni all'obbligo di certificazione verde in zona bianca i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati. Si prevede, inoltre, la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere in zona bianca, tranne che per l'accesso alle predette strutture da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Ulteriori novelle riguardano l'articolo 9-*quater* relativo all'impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto. l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina e per i collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti. Si estende l'obbligo di certificazione verde ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale. Si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale regionale. Si estende l'obbligo di certificazione verde per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esclusi dall'obbligo di certificazione verde sui mezzi di trasporto, oltre ai soggetti esenti, anche i minori di età inferiore a dodici anni. Si stabilisce infine che, per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale, le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi possano essere svolte secondo modalità a campione. del 2021, stabilendo, con decorrenza dal 29 novembre 2021, il principio secondo cui nelle zone gialle e arancioni la fruizione dei servizi e lo svolgimento delle attività e gli spostamenti oggetto di sospensione o di limitazione, in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione contro il Covid-19 o in base a guarigione dal medesimo, oltre che per i minori di età inferiore anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica. Sono esclusi dall'ambito delle nuove norme i servizi di ristorazione svolti all'interno di alberghi o di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati, nonché le mense e i servizi di *catering* continuativo su base contrattuale. L'articolo 6 contiene disposizioni transitorie. Per il periodo che va dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 si prevede che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali nelle zone gialle sono previste limitazioni siano consentiti nelle zone bianche solo ai soggetti in possesso di un certificato verde di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione, nonché ai minori di età inferiore ai dodici e ai soggetti esentati dalla campagna vaccinale. Anche in questo caso sarà sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e *catering* continuativo su base contrattuale. Nell'ambito del capo III, concernente i controlli e le campagne di informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del possesso del possesso delle certificazioni verdi. Tale piano è adottato dal prefetto entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, previa consultazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. I controlli sono effettuati dalle Forze di polizia e dal personale dei Corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, in maniera costante e anche a campione. Si prevede che il prefetto trasmetta al Ministro dell'interno una relazione, con cadenza settimanale, inerente ai controlli effettuati nell'ambito del territorio di competenza. Si dispone altresì che tali attività siano svolte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 8 demanda al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elaborazione di un piano per garantire i più ampi spazi sui mezzi di comunicazione di massa per campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il SARS-CoV-2. L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 101 del 2020, che ha dettato la nuova disciplina per limitare il rischio di esposizione delle persone a livelli anormali di radioattività e di contaminazione dell'ambiente. L'articolo 10, infine, dispone dell'entrata in vigore del presente decreto-legge. Devo dire che, nel corso dell'esame in Commissione, l'obbligo vaccinale è stato esteso, a decorrere dal 15 febbraio, anche agli studenti in corso di laurea impegnati nei tirocini per l'abilitazione alle professioni sanitarie 1.6 (testo 2) e 1.7 (testo 2). Inoltre, è stato specificato che l'esenzione per motivi di salute dalla somministrazione del vaccino possa essere accordata solo dal proprio medico di medicina generale oppure dal medico vaccinatore (emendamento Sono state introdotte poi delle specificazioni per porre rimedio ad alcuni problemi pratici e procedurali che siano riscontrati nella verifica dell'adempimento dell'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario sanitario (emendamenti 1.16, 1.17 e 1.25), anche in conseguenza della scelta del Governo di sostituire interamente il previgente testo dell'articolo 4 del decreto-legge n. 44 del 2021. Sempre in sede di esame in Commissione, l'obbligo vaccinale è stato esteso anche al personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (emendamento 2.9). Sono state poi previste modalità per la verifica dell'adempimento dell'obbligo da parte dei dirigenti scolastici e delle figure equiparate (emendamento 2.18). specificato che la sostituzione temporanea del personale non vaccinato si applica non solo ai docenti, ma anche al personale educativo e ATA (emendamento 2.46). L'emendamento 2.0.4 (testo 3), approvato dalla Commissione, ha previsto per i dipendenti pubblici - e questa è una è una votazione avvenuta soltanto pochi minuti fa - l'assenza giustificata dal lavoro per la somministrazione del vaccino. Nel corso dell'esame in Commissione l'obbligo di possesso del *green pass* è stato espressamente esteso anche ai titolari dei servizi di ristorazione e somministrazione (emendamento 4.28).

è stata introdotta dalla Commissione una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome: delle minoranze linguistiche è stato proposto appunto l'emendamento 9.0.1. Concludo ricordando che, nel corso dell'esame, diversi ordini del giorno sono stati accolti dal Governo con l'impegno ad affrontare in tempi brevi altre rilevanti questioni. soprattutto - e qui voglio sottolinearlo, spero con un minimo di attenzione da parte dei colleghi - l'ordine del giorno G/2463/22/1, votato all'unanimità dalla Commissione, sul tema non più differibile - e qui mi rivolgo anche al presidente Parrini, che ha presieduto egregiamente la Commissione anche allo scopo di venire incontro a questa ormai ormai storica esigenza cui il Parlamento deve dare applicazione - dell'estensione dell'indennizzo per i danni permanenti da vaccinazione obbligatoria anche per quella consistente parte di popolazione per cui non c'è un obbligo, ma solo una raccomandazione. Come è noto, quando c'è obbligo è automatico l'indennizzo, ma sono intervenute sentenze della Corte costituzionale: infatti è previsto per tutti i vaccini obbligatori dalla legge n. 210 del 1992, ma diverse sentenze della Corte costituzionale, lo hanno esteso a vari casi di vaccinazione che invece era solo raccomandata e non obbligata. Non vi sono perciò dubbi sul fatto che la Costituzione imponga di applicarlo anche a questi vaccini; se non lo farà il legislatore, ci penserà la Corte costituzionale. Qualora ciò non dovesse avvenire nell'ambito di un nuovo e imminente provvedimento d'urgenza, come è stato impegnato il Governo - mi rivolgo a tutti i Capigruppo della maggioranza che hanno partecipato a questo tipo di

vi provvederà il Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge n. 221 e n. 229 del 2021, che nel frattempo sono stati assegnati al Senato, in modo particolare alla 1a Commissione affari costituzionali,

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritta a parlare la senatrice Drago. Ne ha facoltà.

in sicurezza di attività economiche e sociali. La relazione illustrativa al decreto recita testualmente: «Il presente decreto mira a proseguire la strategia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19 sul territorio nazionale, basata sul presupposto che la vaccinazione rappresenti un'arma imprescindibile nella lotta alla pandemia, configurandosi come un'irrinunciabile opportunità di protezione individuale e collettiva».

dei tamponi fai da te venduti in farmacia, fece un sorriso sardonico. A distanza di un anno vediamo benissimo qual è la situazione.

La domanda è se ciò non abbia contribuito, rispetto a tutte le altre dinamiche, a impedire il raggiungimento dell'obiettivo indicato nella relazione illustrativa e in premessa. Siamo di fronte a una situazione assurda,

era stato riformulato proprio dalla maggioranza, che prevedeva nel nuovo testo l'esclusione dei tamponi molecolari. Altra parentesi: è sotto gli occhi di tutti il costo elevato di questi tamponi; denuncia una speculazione, che in alcuni casi supera i 150 euro a prestazione. Questo a riprova del fatto che sono interventi che non hanno una loro omogeneità e logicità e tra l'altro si contrastano l'altro si contrastano vicendevolmente. Per quanto riguarda un fatto, che ha dato seguito anche al deposito di petizioni da parte di di alcuni esponenti e comitati delle popolazioni isolane, ho rappresentato una necessità, sottoscrivendo tra l'altro un emendamento della senatrice Angrisani che è stata così gentile da accogliere la mia firma. Anche alcuni senatori di Fratelli d'Italia hanno depositato - mi riferisco a Malan e La Pietra - un emendamento per le isole minori. Che cosa si sta verificando? Nell'imporre questo super *green pass* per tutti i mezzi di trasporto, quindi anche i traghetti, sostanzialmente operiamo una discriminazione nella discriminazione: ovvero, coloro i quali scelgono di non sottoporsi a vaccino, ma in tempi ravvicinati, quindi ogni tre giorni, devono essere

penalizzato, perché con mezzo proprio non avrà la possibilità di attraversare, nel caso della Sicilia lo Stretto, nel caso delle isole Tremiti o altre isole minori chiaramente il mare che li separa dalla terraferma.

evidenziare ed elencare tutte le bugie, le clamorose e pericolose bugie, che questo Governo aveva inanellato sul *green pass*, prima tra tutte la bugia secondo cui il *green pass* e il super *green pass* dovevano servire a creare luoghi di lavoro e ambienti Covid-*free*, dove le persone sarebbero state libere di lavorare e interagire senza rischiare di contagiarsi. Balla pericolosissima, perché ha indotto tantissimi italiani a ritenersi immuni soltanto per avere un certificato e che ha portato alle stelle i contagi, com'è sotto gli occhi di tutti. È stata questa mossa di burocrazia estrema, di bugie e di falsità che ha portato i contagi ai livelli che abbiamo oggi. nonostante l'evidenza e la necessità di stigmatizzare quanto accaduto, non farò questo discorso, perché tutte queste cose ormai sono evidenti a tutti: anche chi ha due o tre dosi si contagia e può contagiare. È molto meno evidente - e quindi merita il mio intervento oggi - ciò che è accaduto in Commissione. Ebbene, in Commissione, con una superficialità che a dir poco questo - con l'importanza e la gravità di un provvedimento che incide così pesantemente sul quotidiano, sulla vita, sul lavoro e sulla salute di tutti gli italiani, con una «soavità» e una noncuranza incredibili, sono stati respinti emendamenti che pure parti importanti di questa maggioranza avevano presentato. avevano presentato. Potrei stare qui tutta la sera, ma vi elenco soltanto quelli che a mio avviso sono i più eclatanti. Il MoVimento 5 Stelle aveva meritoriamente presentato un emendamento in cui

data del 31 marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza, in tutte le parti in cui il decreto-legge prevedeva queste eccezioni alle libertà costituzionalmente garantite. Ebbene, nonostante questa fosse una misura di buonsenso - ovvero

l'emendamento in un ordine del giorno che, come sapete, è un mero auspicio per il futuro. Quindi, questo è stato messo nel cassetto,

stato di emergenza che - lo ricordo - è già stato prorogato sei volte, ben oltre i due anni previsti e, tuttavia, non è andato bene al Governo che si mettesse una fine a tutto questo. Ce n'è anche per la Lega e per il PD, ad esempio: entrambi hanno presentato emendamenti volti a prevedere gli indennizzi in caso di danni da vaccinazione.

il ragazzino, il tredicenne che non è vaccinato, non è guarito e non ha il super *green pass*, anche se deve prendere l'autobus per andare a scuola, non lo può fare, un'ulteriore discriminazione tra quei ragazzi che possono essere accompagnati dai genitori e coloro che invece non possono perché magari i genitori lavorano o perché comunque non hanno un passaggio né i soldi per pagarsi un taxi. Ma no, per loro è impossibile andare a scuola con i mezzi di trasporto. Anche in questo caso, MoVimento 5 Stelle e Italia Viva, che pur meritoriamente avevano previsto emendamenti in tal senso, abbassano le orecchie e dicono: obbedisco.

un nostro emendamento, a prima firma della collega Angrisani e mia, che prevedeva di ripristinare la continuità territoriale con le isole, che oggi è stata interrotta perché chi non ha il super *green pass*,

chi vive in Sardegna o in Sicilia e non può venire in Continente e viceversa. Eppure, anche in questo caso un no immotivato: sardi e siciliani devono per forza essere vaccinati o guariti oppure non si possono muovere dalle isole. Ancora, un altro meritorio emendamento, dell'ottimo senatore Malan, chiedeva che l'Istituto superiore di sanità e l'Istat dessero i dati di mortalità dell'anno appena passato, del 2020, e anche del 2021, in maniera tale da poter confrontare la mortalità generale, per vedere se, confrontando i due anni di pandemia,

per dare una risposta alle tante illazioni, che in questo momento non si fondano su dati statistici reali, ma che circolano e che creano molta apprensione. Illazioni sul fatto che, in quest'anno di vaccinazione spinta, ci siano stati più morti dell'anno scorso. Ebbene, anche in questo caso la risposta è stata che no, non ci deve essere chiarezza, non ci devono essere dati che possano mettere

voi vi assumete una responsabilità. State spaccando il Paese. Non state facendo un'operazione di trasparenza. Non state dicendo le cose come stanno e state ghettizzando una parte di popolazione che, lo ripeto, allo stato non ha obblighi giuridici. La conseguenza qual è? Vi faccio degli esempi concreti. Soltanto oggi, una madre disperata mi ha chiamato dicendomi che, nel primario istituto scolastico della mia città, i ragazzi sono stati chiamati uno per uno dal preside, che ha chiesto loro se erano vaccinati o no. A quelli non vaccinati è stato detto: prendete le vostre cose, chiamate casa e fatevi venire a prendere. Questo perché, essendoci stati due casi di positività, è scattata la norma secondo cui tutti i non vaccinati non possono essere in presenza.

ma nessuno ha scritto che poteva fare il vaccino. È in un limbo e, come lei, vi si trovano tantissime altre persone, non per scelta, che sarebbe comunque accettabile, ma per delle reali situazioni di salute. Ancora, un'altra signora mi ha rappresentato di avere la

come persone di serie B, come bestie. Non valutare attentamente quanto state facendo, con la vostra superficialità, è di una gravità che vi si ritorcerà contro. Signor Presidente, io ho preparato un intervento un po' articolato.

dati parlano chiaro. Noi siamo convinti di essere nella direzione giusta e ringraziamo il Governo per andare avanti in questa strada. È iscritta a parlare la senatrice Garnero Santanché. Ne ha facoltà. oggi noi stiamo parlando di un provvedimento che di per sé è stato superato, perché il Governo ha deciso di fare un regalo agli italiani. infatti il decreto di Natale, poi quello di Capodanno e poi quello dell'Epifania. Questo per dire, in sintesi, che sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico. è diabolico. Il Governo continua nelle sue contraddizioni e vi faccio alcuni esempi, perché credo che debba essere chiara agli italiani la direzione che si sta prendendo.

L'altra contraddizione che vorrei sottolineare in maniera molto chiara è la mancanza di senso del consenso informato. applicato a un trattamento sanitario imposto, per tutte le persone di buon senso e non ideologiche, sia assolutamente irragionevole. Tutti coloro che sono andati a vaccinarsi avuto davanti a sé il modulo recante la dicitura «Acconsento e autorizzo la somministrazione del vaccino». Questa è la formula che si trova in calce al modulo quando si va a fare il vaccino. però evidente che si tratta di un consenso informato presente nei moduli che dà anche la possibilità di rifiutare la somministrazione del vaccino. Il tema, già emerso e che Fratelli d'Italia rileva da molto tempo in maniera evidente, è che oggi si impone con più forza il tema del consenso informato per

Quindi, la domanda che l'Assemblea e i rappresentanti del Governo si dovrebbero porre e che si pongono tutte le persone non ideologiche, ma di buon senso, sia legittimo, ancora oggi, chiedere il consenso di chi è giuridicamente obbligato a fare il vaccino. Secondo noi non perché il consenso informato, anche secondo una recente sentenza della Corte costituzionale, è previsto al fine di garantire la libertà

solo non riguarda il rispetto delle libertà, ma ha anche un effetto sull'imputazione delle responsabilità ed è quello che chiede da sempre il Gruppo Fratelli d'Italia. Se il Governo - non entro nel merito se ha fatto bene o ha fatto male - ha deciso per l'obbligatorietà del vaccino, proprio per essere trasparente e per trasmettere fiducia ai cittadini, se ne dovrebbe assumere tutte le responsabilità,

avere reazioni avverse al vaccino, ma anche per un risarcimento danni. Ricordo infatti - ad esempio - che, se il consenso informato è incompleto e magari - non è detto che sia così - fondato su presupposti scientifici non corretti, c'è anche la possibilità di un risarcimento dei danni. Quindi, il Governo dovrebbe prendere atto che lo scenario è completamente cambiato da quando il vaccino è diventato obbligatorio. C'è dunque un obbligo vaccinale e in questo caso l'obbligatorietà richiede il consenso dell'interessato: per questo diciamo che c'è una contraddizione in termini. Il Governo non solo deve mettere mano immediatamente al consenso informato, ma deve mettere i fondi

che in Europa i casi erano tantissimi e che l'Italia era assolutamente un modello. Colleghi, oggi siete smentiti e forse qualcuno dovrebbe anche

se tutti siamo convinti che il vaccino è utile e dobbiamo convincere ancora i tanti *over* cinquanta che non sono vaccinati, cosa c'è di meglio che dire che il Governo si assume una responsabilità

su questo punto, che è determinante per convincere quegli italiani che ancora non si sono convinti, anche per il susseguirsi di decreti-legge e per la comunicazione che viene fatta, anche da parte della scienza, che critica. Abbiamo sentito il rappresentante dell'OMS che ha detto che certamente non possiamo immaginare di andare avanti con i *booster* ogni tre Colleghi, prendetene atto: le responsabilità si devono far vedere con chiarezza ai cittadini e non c'è strada migliore per convincere gli italiani a vaccinarsi che quella che da sempre propone il Gruppo Fratelli d'Italia. grazie. ieri il numero di decessi nel nostro Paese ha superato quello di tutti gli altri Paesi europei. Credo sia evidente che il super *green* *pass* e ora l'obbligo vaccinale, che tra l'altro sono stati introdotti quando la percentuale di popolazione vaccinata sopra i dodici anni era già prossima al 90 per cento, non siano strumenti utili a contrastare il diffondersi dell'epidemia. Credo che tutti sappiano che nel resto d'Europa l'obbligo vaccinale generalizzato è stato introdotto solo in Austria e Grecia. Continuo a chiedere per quale motivo non siano state utilizzate subito le terapie precoci, sperimentate con successo da medici volontari sin dall'inizio della pandemia. Avremmo dovuto introdurre l'uso della FFP2 per chiunque, dato che sembra proteggere al 98 per cento chi la indossa. Avremmo dovuto utilizzare intensivamente le monoclonali, che rifiutammo nell'ottobre del 2020 quando ci furono offerte gratuitamente 2.000 dosi, per poi acquistarle pochi mesi dopo. Credo, inoltre, che il super *green* *pass* introduca delle restrizioni inaccettabili. Mi riferisco, in particolare, a quella relativa alla circolazione dei non vaccinati sui mezzi di trasporto pubblico e a molte altre attività per cui sarebbero state sufficienti le FFP2. Abbiamo introdotto nel Paese discriminazioni e addirittura una caccia a chi non è vaccinato, che coinvolge purtroppo anche i ragazzi, il cui contagio ha percentuali veramente minime, come se tutti i contagi che si stanno verificando siano responsabilità di una sparuta minoranza. Ci tengo a ribadire di non essere un no vax, ma ritengo debba essere garantita

sempre che ci sia efficacia, e che con la terza dose si ottiene un accettabile grado di protezione, meno efficace contro la trasmissione del virus. Volevate che il CEO della ditta che ha fatto miliardi con il vaccino dicesse che la terza dose non dà protezione? Lo stesso CEO ha immediatamente annunciato che il vaccino contro la variante omicron sarà pronto a marzo, marzo, quando saremo già in un momento in cui i contagi, come negli anni precedenti, diminuiranno e magari, per quando riprenderanno in autunno, si saranno quasi certamente sviluppate altre varianti. Per chi produce vaccini questo è un invito a nozze, come la prospettiva di vaccinare tutta la popolazione ogni quattro o cinque mesi, senza tenere in considerazione che si possono sviluppare malattie autoimmuni e che dopo e che dopo più vaccinazioni si potrebbero abbattere le difese immunitarie. Che la protezione del vaccino sia scarsa lo dicono i contagi in continua crescita e le dichiarazioni di esimi scienziati. Lo dice l'evidenza che anche i vaccinati prendono il Covid, vanno in terapia intensiva e muoiono. Dopo due anni abbiamo dati ancora incompleti e che non permettono un'analisi dettagliata della situazione, dei fattori che l'hanno scatenata e continuano ad alimentarla. Addirittura questa mattina sui quotidiani c'è chi evidenzia come i dati fra i Paesi europei non siano comparabili, perché non vengono presi in modo omogeneo. Sul piano sociale, purtroppo, stiamo riattivando contrasti che non si verificavano da anni e che credo sia estremamente importante non alimentare. Il diritto alla decisione se assumere o meno una qualsiasi sostanza è garantito dalla Costituzione e dalla legislazione europea reso evidente dal fatto che, per essere vaccinati, si continua a esigere una liberatoria firmata dal vaccinato. Ciò avviene malgrado il vaccino non sia innocuo, abbia generato reazioni avverse, alcune delle quali anche letali. È noto come si tratti di un vaccino ancora sperimentale di cui non conosciamo gli effetti a lungo termine che, se si produrranno, ovviamente scaricheremo sulle generazioni future. Credo che la via da seguire sarebbe stata quella tracciata dalla ministra Pisano e recentemente ribadita da Beppe Grillo: si sarebbe dovuto lavorare sul tracciamento e sull'isolamento dei contagiati.

Signor Presidente, l'obbligo vaccinale che è stato introdotto con questo decreto-legge non ha proprio alcun fondamento, né scientifico, né giuridico. E lo sapete benissimo. Non ha un fondamento scientifico, perché nessuno è in grado di dimostrare l'interesse pubblico che si cela dietro questa terapia preventiva; non è in grado di dimostrarlo nessuno, semplicemente perché noi prima del 2024 non avremo i *report* rischi-benefici. Non si può dimostrare scientificamente, ma si può dimostrare invece empiricamente il contrario, visto e considerato che questo presidio terapeutico preventivo è anche sperimentale, proprio perché i *report* rischi-benefici non saranno disponibili prima del 2024. Si può dimostrare in realtà che questo presidio terapeutico lascia circolare i contagi e, quindi, non immunizza. Pertanto, non è in grado assolutamente di garantire alcuna sicurezza, né sui luoghi di lavoro, né sui mezzi di trasporto, né su tutti i luoghi dai quali sono esclusi i non vaccinati. Quindi, il Governo ha creato artificialmente una discriminazione sul piano giuridico che non ha alcun

innumerevole di articoli della Costituzione, a partire dall'articolo 32, ultimo comma, che prevede che la legge non debba superare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; e qua di rispetto della persona umana non se ne vede traccia; secondariamente, il principio dell'inviolabilità della persona umana, all'articolo 2 e, all'articolo 3, anche il principio di pari opportunità, che - come faceva notare anche il senatore Crucioli nel suo intervento - viene violato all'interno delle scuole con le quarantenne differenziate, introducendo per legge una discriminazione infondata - non esiste uno straccio di studio scientifico che la possa supportare - tra studenti vaccinati e non vaccinati; introducendo una discriminazione

per le isole con il *green pass* normale e l'uso delle mascherine FFP2 (la stessa cosa per i mezzi di trasporto e gli studenti), tuttavia dopo è prevista l'introduzione a pieno titolo di questa discriminazione assurda, che fa che fa sì che alcuni cittadini valgano, sotto il profilo dei diritti, meno degli animali - gli animali hanno il diritto a spostarsi, mentre i cittadini non vaccinati non lo hanno - e delle merci. Siamo allo svilimento totale della persona umana. L'obbligo vaccinale per alcune categorie, con la

su cui si fonda la Costituzione. La Costituzione all'articolo 1 prevede questo diritto, in quanto il lavoro fa il discrimine fra una persona libera e una che non lo è. Chi è libero può esercitare democraticamente la sua funzione civica, mentre chi non lo è non può. Quindi, voi avete tolto a quei cittadini i loro diritti civili,

la parità di genere: proprio quelle persone sono le più accanite nella discriminazione di esseri umani che non hanno alcuna ragione fondata per essere discriminati.

questi provvedimenti... PRESIDENTE. Senatrice, qui non c'è nessuno che si deve vergognare. Ognuno esprime la sua opinione. Lei ora la sta esprimendo, e poi sarà il turno degli altri. Non c'è nessuno che si deve vergognare, senatrice.

che doveva essere il baluardo della Costituzione. Ma questa forza politica si è posta a fianco di queste misure, a loro supporto, per opprimere, devastare e cancellare i diritti umani di cittadini italiani che hanno semplicemente fatto la scelta ponderata di non vaccinarsi, di non usare dei prodotti sperimentali sul proprio corpo, cosa della quale hanno pieno diritto: lo dicono lo dicono il Codice di Norimberga, la Convenzione di Oviedo, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Noi, oltre che cittadini italiani, siamo anche cittadini europei l'Europa deve far rispettare le nostre prerogative. L'Europa non può essere semplicemente un contenitore che praticamente produce trattati di natura economica. L'Europa è un contenitore di esseri umani, di persone che hanno dei diritti che devono essere rispettati. I non vaccinati non producono alcun danno ai vaccinati, e questo lo sapete tutti. Le ospedalizzazioni e le terapie intensive sono piene degli uni e degli altri, salvo poi definire non vaccinati i vaccinati con due dosi: chiaramente adesso li avete inseriti nel calderone dei non vaccinati per sbilanciare e giustificare le vostre assurde misure. Ci sono persone ammalate ammalate nelle isole e sono rimaste confinate nei loro territori, impossibilitate ad accompagnare i figli per ricorrere a delle terapie di cui hanno bisogno, oppure a potersi a loro volta curare. Avete ricattato i medici, perché gli avete praticamente imposto, attraverso una serie di restrizioni e ordini professionali, di non

in piedi uno stato di emergenza che si protrae da due anni e vi siete pure permessi il lusso, fuori da ogni limite e paletto costituzionale, di prorogarlo addirittura fino al 31 marzo. marzo. Siamo veramente arrivati a superare tutto quello che non poteva e non doveva essere superato, nel modo più

Sento l'esigenza di intervenire dopo l'ultimo intervento per dire tre cose molto semplici. In primo luogo, è vero che i vaccini non raggiungono il 100 per cento dell'efficacia, ma è anche vero che non abbiamo niente di più efficace dei vaccini in questo momento.

Noi registriamo nel Governo una - chiamiamola così - flessibilità di accompagnamento agli eventi che possiamo considerare frutto di

dobbiamo semplicemente avere quell'atteggiamento di collaborazione di chi sa che sta prendendo delle misure che oggi sono efficaci e che domani potrebbero esserlo meno e richiedere una

Può accadere questo, ma potrebbe accadere anche quest'altro. Cerchiamo, di volta in volta, di intercettare ciò che è meglio per il Paese. Passo alla terza e ultima cosa che voglio dire in questo clima. Ritengo sia un atto dovuto da parte nostra offrire il meglio di ciò di cui disponiamo, con la consapevolezza che stiamo facendo ciò che è possibile. Qualcuno chiede e probabilmente si aspetta che si possa fare l'impossibile. La medicina non fa l'impossibile, ma procede continuamente e costantemente, per prove ed errori, per migliorare sempre ciò che offre.

anche il lavoro della Commissione abbia quell'attenzione e quella capacità di intercettare i problemi del Paese, facendo da ponte tra le regole in stretto senso e il il fenomeno biologico che richiede un diverso approccio anche sul piano comunicativo. Stiamo proponendo un livello di comunicazione eccessivamente incalzante. Stiamo andando incontro a una sorta di obesità informativa che non permette di prendere decisioni serene, lucide e concrete non tanto a chi studia questi fenomeni a chi studia questi fenomeni e problemi, ma probabilmente a chi semplicemente ne raccoglie l'eco attraverso la stampa e i telegiornali. Oggi le persone hanno bisogno di sentirsi più rassicurate a partire - per esempio - da un concetto molto semplice: non basta un tampone positivo per dire che quella persona è malata. Si tratta di due concetti totalmente diversi: la diagnosi di malattia è clinica è clinica e prende in considerazione la persona nella complessità del suo disagio e della sua sofferenza; il tampone positivo è un'allerta, un allarme, e un segnale di prudenza. Se riuscissimo a trasmettere alle persone

Non è così, anche se la soluzione non è ancora così vicina come tutti vorremmo. Stiamo però andando in una direzione che cerca di intercettare i bisogni di salute delle persone e certamente non di danneggiarne la qualità di vita o la vita stessa.

È importante seguire la scienza, perché dà l'*input* per andare avanti. Per questo vorrei ribadire l'importanza fondamentale della vaccinazione come misura per la lotta al virus

Altro punto che vorrei sottolineare, signor Presidente, è la necessità di una maggiore condivisione da parte di tutte le forze politiche dei provvedimenti adottati, di un più costante e continuo confronto con le Regioni e, infine, infine, di una maggiore chiarezza e comprensibilità nel comunicare le misure adottate. Occorrono segnali precisi, senza andamenti ondivaghi, capaci di infondere nei cittadini fiducia e sicurezza. Anche le osservazioni critiche devono essere costruttive e non fuorvianti, per chi già vive conflitti e drammi interiori e nel contesto sociale. Non dimentichiamo mai che la pandemia si vince tutti uniti.

Signor Presidente, la mia sarà una replica breve. Più che altro non starò qui a discutere sui pareri che evidentemente sono di contrasto a questo decreto-legge e agli emendamenti che abbiamo approvato in Commissione e che tra breve saranno posti in votazione anche qui in Aula.

potesse essere quantomeno contenuta nel miglior modo possibile. Certamente l'idea che i certificati verdi possano svolgere un ruolo straordinario, soprattutto per stimolare le persone a concludere il ciclo vaccinale o a vaccinarsi direttamente, mi pare evidente: è una scelta che questo Governo ha adottato, che la maggioranza ha condiviso e che bisogna riconoscere - come più volte ha sottolineato anche il sottosegretario Sileri - è stata presa in considerazione da altri Paesi dopo il nostro, proprio per

il danno che ne può derivare sulla salute del cittadino è minore e, quindi, anche l'impatto sul Sistema sanitario nazionale è molto ridotto; basta confrontare i dati dell'anno scorso con quelli di quest'anno. Con questo decreto-legge si sono poste le basi anche per venire incontro ad altre istanze. È pur vero che l'emendamento non è stato approvato, ma verrà approvato verosimilmente un ordine del giorno molto significativo sul tema degli indennizzi, non solo derivanti - come ho già ricordato - dalla obbligatorietà del vaccino, ma anche dalla raccomandazione dello stesso. In tal senso, devo riconoscere

a una soluzione per fare in modo che i cittadini italiani si sentano comunque tutelati dal nostro Paese e possano quindi essere tenuti in considerazione. Nella mia relazione introduttiva che il tema degli indennizzi è stato tenuto in considerazione in tempi non sospetti, già alcuni anni fa, dalla Corte costituzionale, quando addirittura la Corte era presieduta dall'attuale ministro della giustizia Cartabia. Ebbene, in quella occasione, Corte sentenziò che, anche nei casi in cui non si era in presenza di obbligo vaccinale, vi era la possibilità di concedere

il tema è quello che, in periodo di pandemia, il ruolo del Parlamento sembra affievolito: si opera solo ed esclusivamente con decreti-legge e, quindi, con provvedimenti d'urgenza. il sistema costituzionale bicamerale sembra essere diventato quasi monocamerale, ma in realtà la Camera che viene investita del compito di affrontare, esaminare ed eventualmente migliorare i provvedimenti del Governo lo fa. In questo caso l'ha fatto il Senato. Ritengo, quindi, assolutamente utile essere consapevoli che il ruolo del Parlamento non è affievolito, ma è solo consapevole del momento storico patologico che il Paese sta vivendo.

è per antonomasia l'Aula del confronto; per carità, si possono avere idee differenti - e le abbiamo anche sui vaccini - ma arrivare a paragonare i vaccini, il *green* *pass* e lo stato d'emergenza

saranno vendicati». Quando si usano parole come vendetta, si parla di minacce e di violenza. Non ci stupiamo poi se ci mettiamo a fare finte dichiarazioni a favore dei medici e degli infermieri che rischiano tutti i giorni le violenze e le minacce dei no vax.

Senatrice Ronzulli, la Presidenza si era già riservata la Presidenza si era già riservata l'opportunità di leggere lo stenografico e abbiamo rilevato le stesse parole che lei oggi ha riportato. Pertanto la Presidenza, che aveva già richiamato nel corso del suo intervento la senatrice Granato, sentito il Presidente del Senato, commina la censura, ai sensi dell'articolo 67 del Regolamento.

alle ore 20,35)*. La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del decreto-legge, gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3, 9.0.2, 9.0.3 e 9.0.4. Sono inammissibili, limitatamente alla parte consequenziale che modifica un allegato al DPCM del 2 marzo 2021, gli emendamenti 5.6, 5.9 e 5.10. Sono inoltre improponibili per materia gli ordini del giorno G9.3, G9.4, G9.5 e G9.6 e inammissibili gli ordini del giorno G9.1 e G9.2.

tempo. È un emendamento che chiede l'istituzione di un fondo per l'indennizzo di eventi avversi causati dalla vaccinazione anti-Covid. in Commissione è stato approvato un ordine del giorno in tal senso, firmato dagli esponenti della maggioranza. Noi invece siamo del parere che non dobbiamo chiedere al Governo di approvare una norma; visto che siamo qua

all'articolo 7 è previsto che i prefetti redigano una relazione sull'attività svolta per il controllo dei *green pass* da parte di tutte le Forze dell'ordine, in coordinamento con la polizia locale, e così via.

la relazione venga omessa, perché se c'è un minimo di fiducia nei confronti dei prefetti, forse è meglio lasciarli lavorare anziché fargli produrre carte

svolte a tutela dei cittadini e del rispetto delle leggi, evidenziando in tale ambito qual è l'entità dei controlli di cui al periodo precedente, e cioè il famoso controllo dei *green pass*. Se si corre dietro a tutti i *green pass*, ma lo spaccio di droga continua a essere un mercato libero, l'abusivismo commerciale è in tutte le strade, ivi incluse quelle della Capitale, a pochi passi dai palazzi delle Istituzioni, i *rave party* continuano a tenersi con una tale lassitudine che vengono anche dall'estero a celebrare queste orge di droga e non solo, con stupri e a volte anche omicidi, ebbene sarebbe opportuno tenere presente anche quello, perché il *green pass* non dovrebbe essere l'unico problema.

motivate esplicitamente come tali nelle premesse, e fanno parte di un decreto-legge che, per definizione, deve essere di straordinaria necessità ed urgenza. Non si capisce perché queste e altre norme introdotte dal provvedimento durano spesso fino al 15 giugno, quando

gli eventuali danni derivanti dalle vaccinazioni raccomandate. Ben sappiamo che i vaccini obbligatori prevedono un indennizzo in caso di danni. Con le recenti misure impostate dal Governo si è estesa la platea delle persone

sono coperte dalla legge che prevede un indennizzo. Restano ancora escluse, al momento, le persone che non hanno un obbligo, ma hanno una forte raccomandazione a vaccinarsi. Sardo d'Azione abbiamo portato avanti sin dall'inizio della campagna vaccinale. Più e più volte abbiamo presentato questo emendamento, che purtroppo non ha mai avuto esito. anche in virtù di una sentenza della Corte costituzionale, il resto dei Gruppi parlamentari ha aderito alla nostra iniziativa e, come avete visto, ha apposto tramite il proprio Capogruppo la firma a questo ordine del giorno,

perfezionare la copertura in tempo utile. Quindi rimandiamo al prossimo provvedimento utile, che il Governo prenderà già la prossima settimana: su questo c'è un impegno chiaro da parte del Governo ai massimi livelli. Riteniamo dunque che l'ordine il giorno sia

tra sette giorni. È quindi la strada più breve, che permette di risolvere un problema, attenzionato da tantissimi cittadini. Quindi l'impegno per il Governo è chiaro. L'auspicio è che venga confermato e che venga fatta giustizia per chi fosse danneggiato da un vaccino, che è stato fortemente suggerito e raccomandato dallo Stato.

però ci sono degli ordini del giorno che invece hanno un valore molto più importante di questo modo di dire e questo rientra proprio tra i pochi ordini del giorno che debbono essere ascoltati e soprattutto attuati. Nel dispositivo non c'è scritto: «a valutare»,

È dovere di questo Parlamento e del Senato agire per una norma specifica su questo. È un dovere; non è un emendamento o un ordine giorno come gli altri. gli altri. Invito i colleghi a mantenere la comunità di intenti trovato in Commissione, ad approvare questo ordine del giorno e al prossimo provvedimento, come dice

prevede la Costituzione, noi siamo altrettanto un organo costituzionale e abbiamo il dovere di legiferare su questo. Non possiamo rimanere bloccati da una

lavoro che per primo ha svolto per coordinare e portare a questo risultato. Tutti avremmo voluto l'approvazione degli emendamenti e, quindi, di una norma precisa nella conversione del decreto, ma l'impegno

Ringraziamo tutta la Commissione per il lavoro svolto e per aver dato al Parlamento la sua giusta collocazione in termini di sostegno ai cittadini, a qualsiasi cittadino, in questo caso specifico per quanto riguarda la garanzia dell'impegno del Governo, in tempi ben precisi, a garantire indennizzi a chi ha dovuto subire delle invalidità permanenti proprio a causa del vaccino. È una bella pagina che la maggioranza ha scritto e di conseguenza siamo certi che il Governo non si sottrarrà poi all'impegno che oggi prende con questo Parlamento e con tutti i cittadini.

favorevolmente. Il Parlamento invece, non si sa perché, si è piegato al *Diktat* del Governo. Ora si dice che si è preso l'impegno e che si poteva votare subito; per questo io non potrò votarlo favorevolmente, pur condividendo nel merito l'iniziativa, e mi asterrò.

2.29, 2.30, 2.32, 2.33, 2.45,

umano, fate un pensierino su queste persone che stanno subendo delle conseguenze gravi sul piano della salute per un vaccino sperimentale che avete imposto con l'obbligo.

era molto pericolosa e sappiamo bene quanti morti ci sono stati in particolare in quell'area, con una mortalità che arrivava anche al 7-10 per cento dei contagiati. Queste sono le condizioni in cui questo maresciallo ha lavorato. Poiché in quel periodo ha contratto la malattia, dalla quale è guarito, egli ha ritenuto di non rivaccinarsi in questo periodo e, di conseguenza, è stato sospeso dal servizio. quadro. L'emendamento 2.29, a prima firma della senatrice Rauti, e gli altri a prima firma del senatore Iannone e a mia prima firma vanno nella stessa direzione. Se l'obbligo vaccinale per le Forze di polizia e per le altre categorie per le quali è previsto

ma che se si vaccinano non ci sono i soldi. Veramente qui andiamo oltre ogni limite di logica e, francamente, anche di elementare umanità.

in origine richiedeva che per alcune categorie di lavoratori pubblici - quelli delle funzioni centrali - venisse concessa una giornata di permesso per poter andare a fare il vaccino. In una prima riformulazione tale permesso è stato esteso a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e nella terza riformulazione, su nostra richiesta, anche al settore privato. accolto la riformulazione e ha dato parere favorevole alla proposta di consentire il giorno di permesso in modo equanime ai lavoratori del settore pubblico e di quello privato. Purtroppo, poi, come spesso accade in fase di esame in Commissione bilancio, MEF, Ragioneria generale e quant'altro, soliti problemi di copertura e si è ritornati a una versione precedente. Ben venga - ci mancherebbe - è ottima cosa che venga concesso ai dipendenti pubblici di esercitare il loro dovere-diritto di vaccinarsi, però non vogliamo che si crei una disparità. Con l'approvazione di questo emendamento avremo lavoratori nel privato con obbligo vaccinale che per vaccinarsi dovranno prendere un giorno di ferie qualora non riuscissero a trovare uno *slot* disponibile di domenica o nel loro giorno di riposo, e

ingiusta. Vorremmo un trattamento identico per i lavoratori del pubblico e per quelli del privato. Se non è possibile, preferiamo che vi sia un'uguaglianza, purtroppo, al ribasso: non vogliamo figli e figliastri,

potrà fruire della possibilità di andare a vaccinarsi senza che per questo si perda un giorno di lavoro. Speriamo sempre e stimoliamo il Governo a trovare le risorse in un secondo momento, al più presto, affinché questa possibilità possa essere estesa ovviamente anche ai lavoratori del settore privato.

4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15,

cioè quella relativa agli abitanti delle isole, che sono doppiamente discriminati rispetto ad altri concittadini italiani che decidono di non vaccinarsi, ma che possono

di un trattamento equo per i cittadini delle isole.

in dichiarazione di voto su questo emendamento a prima firma del senatore La Pietra, che chiede l'esenzione per i soli residenti delle piccole isole in ambito regionale. Qui abbiamo degli effetti paradossali, che sono già stati illustrati, di persone che non possono andare in ospedale, perché non hanno il *green pass*. Ci sono delle isole in cui addirittura non c'è neanche un posto per fare il tampone, all'interno dell'isola, e quindi gli abitanti devono prendere un mezzo pubblico per andare in un'altra isola o per andare sul Continente, sulla terraferma. Ci sono addirittura casi di persone che vorrebbero fare il vaccino, ma non possono prendere il traghetto per andare a fare il vaccino, perché non hanno fatto il vaccino. Sono questioni paradossali, che meriterebbero una certa attenzione, perché riguarda persone reali.

Quindi, io sto terminando l'articolo 4 e lo devo mettere in votazione. Mi deve dare gentilmente il parere

aggiuntivo 5.0.6 (testo 2) che la Presidenza ritiene proponibile solo se riferito all'articolo 4.

Parente e su cui ci eravamo fermati prima, in realtà è stato votato dalla Commissione e dovrebbe essere indicato come della Commissione. È quello che ha creato il *misunderstanding* con il relatore, che chiaramente non se lo è visto segnato come ordine del giorno della Commissione. Poi vi sono altri ordini giorni mancanti all'articolo 5.

L'emendamento 5.0.6, che lei adesso sta spostando all'articolo 4, è stato bocciato dalla Commissione (è il tema, ben noto, delle parafarmacie). Adesso lei lo rimette in votazione; ma a me risultava in fase di ritiro. Così era l'impegno; credo Io non l'ho ritirato e facevo riferimento alla proponibilità. Mi scusi, ma il relatore mi ha detto che è favorevole. Io qui ho letto, dalla Presidenza, che l'emendamento 5.0.6 (testo 2) (già è proponibile a condizione che sia riferito all'articolo 4. io sto gestendo tecnicamente il fascicolo. Questo emendamento lo propongo ora all'articolo 4; altrimenti, secondo le indicazioni della Presidenza, per me non è più

sono comunque oggi al voto in Aula. Allora, aspettate, sul parere contrario del relatore voglio il parere del Governo. 5.0.6 aveva parere favorevole del Governo;

la condizione di improponibilità che è stata posta dalla Presidenza, se fosse rimasto all'articolo 5. Io so bene quello che è accaduto in Commissione. So bene che vi erano i pareri favorevoli sia del Governo che del relatore,

quest'ultimo poteva procedere verso la possibilità compiuta di applicare questo indirizzo, che in qualche modo è stato dato attraverso la riformulazione del Governo.

provato anche a trovare una formulazione, vorrei chiedere al suo rappresentante se ci può essere un impegno per fare in modo che questa operazione possa andare avanti nell'interesse dei cittadini.

chiediamo una sospensione e una riunione di maggioranza perché non sono stati rispettati gli accordi.

Per parte nostra, come già avevamo detto e come hanno già fatto i colleghi del MoVimento 5 Stelle, che ringrazio - hanno la nostra stessa identica posizione, sostenuta anche dai colleghi e dalle colleghe del PD

Signor Presidente, proprio oggi credo di aver letto sui giornali che è stata approvata alla Camera una legge, a prima firma Francesco Silvestri, esponente del MoVimento 5 Stelle, che cerca di normare in qualche modo l'attività delle lobby di Camera e Senato. credo che la dialettica che si sta svolgendo su questo emendamento non possa essere limitata a un discorso di lobby, ma debba essere elevata a un discorso di buonsenso.

non credo un chirurgo di fama internazionale - svolge l'operazione di inserire un bastoncino all'interno del setto nasale dei pazienti. Ebbene, credo che questa operazione semplicissima, a un costo abbastanza basso (15 euro), possa essere effettuata sia nelle farmacie che nelle parafarmacie.

del virus *(Applausi)* e dai costi da sostenere, almeno evitiamo il disagio quotidiano - alle famiglie, ai bambini e agli anziani - di dover fare file chilometriche presso un solo centro all'interno dei paesi. Mi sembra una misura che tutti possiamo condividere. Prego il Governo,

Signor Presidente, credo che la saggezza del senatore Errani sia riconosciuta da tutti i componenti di quest'Assemblea. Mi associo alla sua richiesta e attendo un impegno preciso del Governo, anche perché noi gli impegni - lo dico soprattutto al centrodestra e a Italia Viva - li rispettiamo.

con il centrodestra e Italia Viva che hanno mandato sotto il Governo in Commissione. Assumiamo questo atto di responsabilità, ma lo chiediamo anche con un intervento in Aula al Governo. Dispiace, e

la salute*. Ringrazio il senatore Errani perché ha indicato una via mediana e, quando c'è una via mediana, è più facile per ognuno di noi raggiungere la destinazione.

Presidente, credo di aver dato un messaggio molto chiaro, ovvero quello di evitare divisione e di seguire una via mediana.

Colleghi, siamo sufficientemente adulti. Se ho l'indicazione della prima firmataria dell'emendamento, che mi corregge nella mia la sua volontà è la trasformazione in ordine del giorno, io debbo rispettare la volontà del

vorrei chiarire ai colleghi che per noi l'ordine del giorno non è l'emendamento. L'ordine del giorno è l'impegno nei termini in cui l'ha preso il Governo in quest'Aula.

Signor Presidente, è molto apprezzabile lo sforzo di mediazione che viene sia dal senatore Errani sia dal Governo. Ora, però, il senatore Errani ha specificato che l'ordine del giorno non è il contenuto dell'emendamento.

facilita quella che è diventata una moda, ma che certamente non va bene, e cioè fare troppi tamponi. I tamponi, in questa fase, non vogliono dire quasi nulla, perché

a prendere in considerazione le problematiche che sono state portate avanti, questa Aula lo può votare all'unanimità. Se, invece, il testo dell'ordine del giorno è la ripresa del contenuto dell'emendamento, evidentemente c'è un contrasto di fondo, che è legittimo. Quindi, non è una via mediana, ma è una via confusa, perché si prende il contenuto di un emendamento su cui c'è stato una bocciatura e lo si mette all'interno di un ordine del giorno. Signor Presidente, vorremmo pertanto il contenuto dell'ordine del giorno è molto chiaro e non ci sono equivoci.

dall'emendamento - cioè dal fatto che noi abbiamo un problema di pressione molto forte in questo momento da parte dei cittadini per quanto riguarda i tamponi

il Governo, vista la situazione di pressione molto forte e di sofferenza dei cittadini per quanto riguarda la possibilità di poter effettuare

Chiederò alla senatrice De Petris un testo scritto, perché le sottoscrizioni sono da parte del MoVimento 5 Stelle e da parte del PD.

Ci sono cioè degli emendamenti trasformati in ordini del giorno che, nel fascicolo, mancano.

Ci sono comunque degli ordini del giorno approvati, che devono essere presenti nel fascicolo, come Commissione. PRESIDENTE. Accolti o approvati?

Sono stati approvati e sono quelli che compaiono anche nel fascicolo per l'Assemblea. Quelli che sono stati accolti in Commissione non vengono riproposti in Assemblea. Siamo tutti colleghi e seguiamo tutti le stesse procedure.

alcuni articoli e per altri no.

esauriscono la loro vita in quel momento, in Commissione. Soltanto quelli che vengono ripresentati per l'Assemblea vengono sottoposti al voto dell'Assemblea. Quindi, il mistero è facilmente chiarito.

preoccupazione da parte della senatrice Parente, vorrei provare a rassicurarla con parole chiare. Il fatto che l'ordine del giorno sia stato oggetto di un parere favorevole e di un accoglimento in Commissione significa, in termini procedurali, che l'Aula non si pronuncia nuovamente su quell'ordine del giorno, e cioè nuovamente non viene alla sua attenzione. Termina la sua vita in questo senso, ma il significato politico non termina, perché ci sono stati in Commissione un accoglimento e un parere favorevole del Governo. Quindi, la senatrice Parente deve sentirsi lieta del fatto che la sua posizione è stata accolta dal Parlamento.

Presidente Parrini, io le ridò la parola e spero che sia chiarificatrice di qualunque dubbio, al fine di poter andare avanti. Ne la potenza chiarificatrice delle mie parole purtroppo non dipende soltanto dalle mie parole. *(Applausi)*. Allora, provo a ridirlo. In Commissione ci sono stati degli ordini del giorno che hanno ricevuto un parere favorevole del Governo e sono stati accolti. Quindi, c'è stata politicamente una decisione di condivisione del contenuto di quegli ordini del giorno,

o che, pure accolti, sono stati ripresentati per l'Aula, vengono all'esame e all'attenzione dell'Aula. Non c'è alcuna incongruenza e soprattutto vorrei dire che non ci sono ordini del giorno di serie A o di serie B, a seconda che vengano o non vengano esaminati in Aula. Gli ordini del giorno sono di serie A o di serie B a seconda che vengano o meno condivisi. Quindi, tutti quelli condivisi sono figli allo stesso titolo della stessa approvazione e condivisione.

bianche in zone gialle è l'unico punto che il nostro movimento, anche in sede di Governo, non ha pienamente condiviso. I nostri tre Ministri hanno espresso una riserva, quindi il nostro emendamento è conseguente. votare questo emendamento soppressivo, perché riteniamo che... vado avanti ugualmente, grazie per l'aiuto. sminuire l'azione del Governo e a renderla inefficace, perché l'azione del Governo è stata meritoria nell'individuare delle zone colorate (le famose Regioni gialle, bianche, arancioni, rosse e via dicendo), e i cittadini hanno imparato a regolarsi di conseguenza. Quindi un comportamento corretto da parte della cittadinanza ottiene una risultanza premiale. Se il Governo con questo articolo 6 temporaneamente decide di sopprimere la situazione premiale - mi si conceda questo termine un po' particolare viene meno l'attenzione del cittadino a tenere un comportamento consono, perché capisce che non c'è più una logica di bastone e carota, ma solo di bastone e bastone. Quindi è indifferente l'attenzione da parte del cittadino. In quest'ottica, proprio per non smentire la linea politica del Governo, riteniamo che l'articolo 6 sia sbagliato e manteniamo l'emendamento soppressivo.

Se è la versione riformulata, è un errore che sia qua, o comunque va votata; se è la vecchia versione, è ovvio che va ritirata. Se è la vecchia versione, come è stato detto, è stata riformulata. Questo è quello che mi ha detto il relatore. È per questo che faccio riferimento ai proponenti, che sapranno se è la versione originale o riformulata.

Gli ordini del giorno accolti in Commissione sono accolti, punto. Quello del senatore Rufa, salvo che non sia un altro ordine del giorno (e non lo è, perché è la versione vecchia non riformulata), dovrebbe essere stato ritirato e quindi non va votato, né altro.

È evidente che, così com'è stato approfondito in Commissione, i Carabinieri forestali sono agenti di pubblica sicurezza. Il punto non è questo, quanto quello che fra le funzioni ordinarie assegnate al Corpo non vi è quella del controllo dell'ordine pubblico generalizzato. Al di là di quanto disposto dalla circolare, alcuni comandanti regionali e il Comando generale avevano sollevato la possibilità di impiegare o meno, a legge vigente,

inserendo e citando espressamente i componenti del Corpo forestale, era volto a dare una copertura a questi agenti delle nostre Forze dell'ordine nei servizi che chiediamo loro di applicare. Quindi, al di là della parte della copertura già prevista, ritiro l'emendamento - ci mancherebbe - ma chiedo al Governo di verificare che quei servitori dello Stato stiano svolgendo quelle funzioni in tranquillità per tutti, perché diversamente sarebbe un problema. Noi facciamo uno sforzo in più, assegnandoli a un compito diverso; facciamo in modo che possano farlo in sicurezza per i cittadini e per loro stessi.

Visto il tema posto con l'emendamento 5.0.6 (testo 2), si impegna il Governo «a individuare le soluzioni più adeguate per assicurare la più ampia disponibilità per l'accesso dei cittadini alla fruizione di tamponi antigenici».

Il virus, purtroppo, ci ha abituati a trattare l'epidemia per fasi, e questa è una fase in cui, data la recrudescenza dei contagi e l'arrivo di una nuova variante, siamo costretti a prendere provvedimenti, da una parte, di contenimento dell'epidemia, e dall'altro, di cambiamento di approccio all'epidemia Molti scienziati del mondo ci dicono che questo può essere l'inizio dell'endemizzazione dell'epidemia; è molto probabile. Credo

nell'alveo dell'impalcatura legislativa che abbiamo, e mi riferisco all'emendamento sulla questione dei tamponi. Ribadisco che mi spiace molto dover constatare che sono state usate parole pesanti in alcune dichiarazioni pubbliche. scritto del mio intervento e chiederei anche a chi fa talune dichiarazioni pubbliche di avere un confronto sui temi che abbiamo affrontato.

Fratelli d'Italia, ovviamente, voterà contro questo provvedimento, per una serie di circostanze che attengono al metodo, che possiamo

Per quanto riguarda il merito, dobbiamo purtroppo constatare che ancora si insiste sui provvedimenti coercitivi e, invece, non si adottano i provvedimenti di contenimento sanitario. Non li spiego, ma, per esempio, collega Sileri, sono la ventilazione forzata nelle aule scolastiche, il potenziamento dei trasporti, le terapie domiciliari, l'aggiornamento dei vaccini (perché ormai anche l'OMS ha detto che con i vaccini vecchi è inutile continuare a vaccinare), il tracciamento (che noi abbiamo perso completamente) il sequenziamento (ancora più importante, che noi non stiamo facendo in misura sufficiente). Non siamo riusciti a coinvolgere ancora i medici di medicina generale sulla necessità di arrivare a vaccinare i sei milioni di italiani che ancora non si sono vaccinati. Dovremmo valutare attentamente la vicenda dello *screening* anticorpale. Ricordo che la Svizzera adottato questa metodologia per rilasciare addirittura un documento come il *green pass*. Rispetto a tutte queste inadempienze, è del tutto evidente che non possiamo continuare a operare coercizioni delle libertà individuali e delle libertà di impresa. Questa non è un'attenuante generica del fatto di non riuscire ad adottare i provvedimenti sanitari, che invece sono necessari. Concludo con una battuta. Siamo rimasti impegnati, per una giornata, un pomeriggio e una nottata, per convertire un decreto-legge morto, perché ogni provvedimento è stato superato dai tre successivi decreti. abbiamo iniziato il 2022 in modo tragico, per quello che riguarda il procedere dei lavori parlamentari. Faccio appello alla Presidenza, perché non si ripeta quello che sta accadendo e quello che è accaduto oggi. *(Applausi)*.

visto il contesto, visto l'orario e viste le condizioni, penso anche che il lavoro che abbiamo fatto oggi sia importante. Siamo stati tante ore in Commissione e anche il dibattito, per quanto acceso, svolto in Aula ha dimostrato la ricchezza del dibattito in Commissione

a quello che hanno detto il presidente Draghi e il ministro Speranza l'altro giorno, l'avversario da battere in questo momento sono i no vax. Conosciamo la situazione epidemiologica e i numeri paurosi di questi ultimi giorni, tra contagi e morti; oggi abbiamo il numero più alto di deceduti di questa quarta ondata.

poter migliorare l'uso dei tamponi da parte dei cittadini. Sappiamo che ci sono code lunghissime davanti alle farmacie. L'unica questione che mi preme sollevare, perché ancora una volta è il nostro punto di vista come Gruppo Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali, è quello della diseguaglianza dei vaccini nel mondo. Pensiamo soltanto agli 800 milioni di persone che sono prive di energia elettrica nel mondo. È un dato che ci deve far riflettere, perché certamente dalla pandemia finiremo nell'endemia, ma quando?

con convinzione. Forza Italia era anche per l'obbligo vaccinale, così magari si sarebbero risolte tante cose. *(Applausi)*. Con il provvedimento è stato assolutamente fatto in modo che ci fosse meno pressione sui reparti ospedalieri. Forse infatti qualcuno in quest'Aula non ha ancora capito che c'è una pandemia. Quando sento parlare di scienza, sarebbe meglio che parlassero tutti di calcio, così almeno non ci sarebbero delle cose da fare. Credo che il maggiore diritto sia quello alla salute,

vaccinati. Ho sentito fare l'esempio della Gran Bretagna. Vorrei solo dire una cosa in favore del nostro sistema sanitario. Certamente in Gran Bretagna non ci sono tracciamenti, non ci sono tamponi, ma non ci sono neanche i numeri reali. Un test molecolare

Tengo a ricordare che la posizione della Lega si esprime con i voti ufficiali, come in questa occasione.

lo fa, come ribadito più volte, solo per evitare la promulgazione di norme inutili e vessatorie, che non hanno effetto alcuno sul quadro sanitario, ma che potrebbero produrre solo esasperazione È un tema che non va sottovalutato e ne sono un chiaro esempio le minacce provenienti dall'ala estrema della galassia no vax, espresse con invio di proiettili al presidente del Trentino-Alto Adige, Maurizio Fugatti, e con gli insulti *social* al

Il secondo appunto è che non bastano i vaccini: sono l'azione primaria e principale di lotta al Covid, ma va ribadito che anche i vaccinati si contagiano e possono contagiare. Quindi va messa in campo tutta un'altra serie di azioni di lotta al Covid. Concludo dicendo che, seppure in questi mesi non sono state disposte chiusure di esercizi commerciali e di attività di natura economica, la sostanza della realtà, come abbiamo visto tutti durante il periodo della pausa natalizia, è che tantissime attività erano comunque chiuse o lavoravano al 10 per cento. Tutte le restrizioni collegate al *green pass* base o al *green pass* rafforzato, o semplicemente la paura che i cittadini avevano di spostarsi, hanno portato ad un annullamento delle entrate. Concludo dicendo che questo annullamento delle entrate, simile, se non uguale, alle chiusure imposte da un *lockdown*, deve comportare il prima possibile l'approvazione in Consiglio dei ministri di un sostanzioso decreto ristori, a favore di famiglie e attività economiche. *(Applausi)*. Detto questo, voteremo favorevolmente. *(Applausi)*.

a Roma e a Milano: c'è un pezzo di Paese che vuole andare in piazza. È un pezzo di Paese che ha onorato il Paese stesso ed è importante sottolineare questa manifestazione e questo dissenso che c'è. Sono contento anche del fatto che Italexit porterà a Milano il premio Nobel Montagnier. Quella che avete intrapreso è una strada che esclude, che discrimina e che ormai è persino fuori fuoco. L'emergenza sanitaria l'avete trasformata in una emergenza burocratica

esprimerà delle idee che non vi piacciono. Qui dentro siete ormai una maggioranza larghissima, ma provate ad ascoltare questo Paese, perché non è così lunare e non è così marziano. Imparate a prestare ascolto a chi oggi dissente.